da loro ritenuto iniquo e lesivo dell'immagine dell'Italia e delle Forze dell'ordine, con cui il capo della Polizia *pro tempore*, Alessandro Pansa, ha disposto nel marzo 2014 una notevole riduzione della sanzione disciplinare inflitta all'assistente capo della Polizia, Massimo Nucera, per le false dichiarazioni rese in relazione all'irruzione nella scuola Diaz nella notte del 21 luglio 2001, durante il G8 di Genova. Ai fini della risposta, ritengo utile ripercorrere brevemente le vicende processuali e disciplinari che hanno interessato il signor Nucera a seguito dell'operazione di polizia appena citata. È utile mettere a disposizione il quadro d'insieme delle sanzioni penali e disciplinari irrogate all'assistente capo per la condotta tenuta in occasione dei fatti del G8, evidenziando tra l'altro che la sanzione richiamata nell'interrogazione non è stata l'unica sanzione disciplinare adottata nei confronti dell'assistente capo. Il signor Nucera, in primo grado, è stato assolto dalle imputazioni di falso ideologico e calunnia aggravata, mentre nel giudizio di secondo grado la Corte d'appello di Genova l'ha condannato per il primo dei due reati a tre anni e otto mesi di reclusione, condonati nella misura di tre anni per effetto dell'indulto e, in aggiunta, alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. Per il reato di calunnia, invece, la stessa Corte d'appello ha dichiarato la prescrizione. Il procedimento penale è proseguito davanti alla Corte di cassazione che, nel luglio 2012, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena inflitta per il reato di falso, rideterminando la condanna in tre anni e cinque mesi di reclusione, condonati - come detto - nella misura di tre anni, ferma restando l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. A seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il capo della Polizia ha disposto, con provvedimento del 9 luglio 2012, l'immediata sospensione del signor Nucera dalla qualifica per tutta la durata della pena principale ed accessoria e, quindi, per un totale di cinque anni e cinque mesi. Per i medesimi fatti definiti in sede penale, sono state promosse nei confronti del signor Nucera due distinte azioni disciplinari. La prima, che è quella a cui fanno riferimento gli interroganti, si è conclusa con un provvedimento che il capo della Polizia, nell'esercizio dei poteri discrezionali conferitigli dalla legge, ha emesso a seguito di una valutazione complessiva della posizione dell'interessato. La seconda azione disciplinare è stata promossa nei confronti del signor Nucera nella sua qualità di agente di polizia giudiziaria, su iniziativa del procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova. Nel maggio 2015, al termine della prima fase del procedimento, la commissione di disciplina istituita presso la predetta Corte d'appello ha inflitto la sospensione dall'impiego per

a conclusione della quale ricordo che il signor Nucera è tuttora sospeso dal servizio, con relativa decurtazione della retribuzione mensile,

ricordiamo tutti la ferita che ha costituito per l'onore delle Forze dell'ordine, per l'onore della nostra Repubblica, il comportamento tenuto nella scuola Diaz di Genova. Ciò che è successo è di una gravità enorme ed è soprattutto rilevabile da coloro che hanno stima, come noi, delle Forze dell'ordine e del modo in cui, di norma, espletano il proprio dovere. Il signor Nucera ha percorso una serie di provvedimenti giudiziari e disciplinari ed ha avuto la fortuna di beneficiare dell'indulto e della prescrizione per parte delle pene che dovrebbe effettivamente Questo non è avvenuto. Lei ha fatto riferimento, nella sua risposta, all'esercizio del potere discrezionale del capo della Polizia. Noi proprio a quello facciamo riferimento. la pena amministrativa inflitta dalla commissione - ci pare, in questo caso, cozzi in modo netto con il sentire comune di tutti quelli che conoscono i fatti di Genova. Oltre tutto parliamo di una persona che, dal comportamento e dalle decisioni, non appare pentito di quanto è avvenuto, della sua partecipazione a quei fatti. Per questo non posso dirmi soddisfatto:

Signor Presidente, il senatore Campanella lamenta la mancata presentazione, da parte del sindaco di Bagheria, della relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta, prescritta dall'articolo 17 della legge regionale siciliana n. 7 del 1992. In relazione a tale inadempienza, chiede al Ministero dell'interno di sollecitare il competente assessorato della Regione Siciliana alla tempestiva applicazione della norma dettata dalla legge regionale siciliana n. 48 del 1991, che prevede la rimozione o sospensione di amministratori nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge. Va innanzi tutto sottolineato che le iniziative finalizzate a promuovere la rimozione del sindaco di Bagheria, per le motivazioni indicate nell'interrogazione, sono riservate alla stretta competenza dell'amministrazione regionale. Ciò detto, va anche rappresentato che il 5 aprile scorso l'assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana ha effettuato una indagine ispettiva nei confronti del Comune di Bagheria al fine di verificare, tra l'altro, la circostanza relativa alla mancata presentazione da parte del Sindaco della citata relazione scritta. Dagli accertamenti svolti è effettivamente emerso che dalla data dell'insediamento del primo cittadino, risalente al giugno del 2014, alla data dell'ispezione, l'adempimento non risultava essere stato effettuato. Il predetto assessorato ha riferito anche quanto affermato dall'amministrazione comunale in merito alla vicenda, e cioè che il ritardo nella presentazione della relazione sarebbe stato determinato dalla mole di lavoro, ordinario e straordinario, connesso allo stato di dissesto dell'ente locale, nonché dalla necessità di predisporre tutti gli atti richiesti dall'organismo straordinario di liquidazione. Sempre secondo l'amministrazione comunale, l'inottemperanza all'obbligo di legge sarebbe inoltre dipesa dalla rimodulazione dell'apparato amministrativo interno al Comune, oggetto di una ridefinizione nell'ottica di una razionalizzazione delle spese conseguente allo stato di dissesto dell'ente locale. Quanto agli sviluppi più recenti della vicenda, informo che il 5 settembre scorso l'assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica ha formalmente diffidato il sindaco a presentare la relazione in questione, avvertendo che l'inosservanza dell'adempimento è rilevante ai fini dell'avvio del procedimento di rimozione dall'incarico. Contestualmente l'assessore ha disposto, tramite l'ufficio ispettivo competente, un monitoraggio periodico dell'andamento dell'esercizio delle funzioni del sindaco nella materia in questione. Il 29 settembre, il sindaco di Bagheria, in risposta alla diffida, ha comunicato all'assessore regionale di aver inviato la relazione in questione, relativa ai periodi 2014-2015 e 2015-2016, al Presidente del Consiglio comunale per il seguito di competenza. Questo è quanto è risultato dall'attività istruttoria svolta dagli uffici del Viminale.

2015: il tempo non è indifferente in questi atti, anche perché nel tempo si possono venire a creare condizioni di sostanziale disconoscimento della legge. Mi spiego: la mia interrogazione consegue a una serie di interrogazioni presentate e di tentativi di accesso agli atti, posti in essere da due consiglieri del Comune di Bagheria,

deve poter porre in atto nei confronti dell'Esecutivo, in questo caso il sindaco. Sorvolando ora sul caso specifico

di funzionamento del controllo da parte dell'assessorato, che si è attivato con tempi suoi (parliamo di segnalazioni fatte nell'arco di un anno).

relazione - come il sindaco ha comunicato e non ho motivo di dubitarne - è stata ora trasmessa al Presidente (che è dello stesso partito del sindaco),

questa richiesta è stata reiterata e i controlli vengono effettuati *de visu*, e nessuna risposta è ancora stata data. stata data. Ci troviamo quindi di fronte a delle criticità operative, perché noi esercitiamo un controllo comunque distante, atteso che il primo controllo avviene da parte della Regione. Quest'ultima, per motivi che non mi è dato conoscere, ha un atteggiamento di inerzia, spero non di omissione: siamo in bilico tra i due termini. Noi ci ritroviamo di fronte alla necessità di un controllo che deve poter essere effettuato, anche per dare delle risposte politiche al territorio, ma che di fatto non viene posto in essere. Per cui spero e conto, conoscendo la sua diligenza, che ci sia un prosieguo nell'azione di sollecitazione nei confronti dell'amministrazione della Regione siciliana, in modo tale che il giusto diritto dei cittadini ad essere informati sull'operato della propria amministrazione abbia un soddisfacimento adeguato.

Signor Presidente, il senatore Malan esprime critiche sull'operato della questura di Prato in occasione dei servizi di ordine pubblico predisposti per la visita del Presidente del Consiglio dei ministri avvenuta nel capoluogo di quella provincia lo scorso 24 settembre. In particolare, egli lamenta che la rimozione parziale di uno striscione di netta disapprovazione dell'azione del Governo, affisso dal coordinamento provinciale giovanile di Forza Italia a pochi metri da un luogo dove il Presidente del Consiglio dei ministri si sarebbe recato il giorno successivo per un'iniziativa pubblica, avrebbe determinato una violazione della libertà di manifestazione del pensiero. Come già rappresentato dal Ministro dell'interno in una recente seduta di *question time* alla Camera, l'episodio è stato evidentemente il frutto di una valutazione prudenziale compiuta nell'ambito degli scrupolosi e mirati servizi di vigilanza, osservazione e prevenzione attivati nella zona del museo Pecci, teatro della visita istituzionale del Presidente del Consiglio; valutazione prudenziale volta ad evitare che l'esposizione dello striscione in una posizione di estrema evidenza, pur costituendo libera espressione di dissenso, potesse dare luogo a turbative dell'ordine pubblico. La decisione del personale della locale questura di rimuovere parzialmente lo striscione va interpretata da tale angolo visuale e ad essa non va attribuito alcun intento censorio. Peraltro, il predetto personale, nella logica di un dialogo civile, ha cercato di contattare gli autori dello striscione per invitarli a rimuoverlo, senza tuttavia riuscirvi, in quanto non erano presenti *in loco*. Per cui, nel dare atto che lo striscione non conteneva frasi offensive o minacciose e che quanto espresso in esso rientrava in una cornice di libera e legittima manifestazione del pensiero, che deve essere sempre consentita, tuttavia che il comportamento, anche dialogante, delle Forze dell'ordine sia stato mirato esclusivamente a rimuovere ogni ostacolo alla ordinata riuscita dell'evento. Su un piano più generale, la vicenda costituisce l'ulteriore riprova che l'attività delle Forze di polizia impegnate nei servizi di ordine pubblico presenta profili di notevole delicatezza, dovendo realizzare un equo contemperamento tra la garanzia dei diritti costituzionali di riunione e manifestazione del pensiero e l'esigenza del mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. La difficoltà del compito scaturisce anche dal fatto che tali tipi di servizi richiedono spesso valutazioni e decisioni non semplici in scenari connotati da criticità operative. Comunque, assicuro che le Forze di polizia continueranno a svolgere, a Prato come nel resto del territorio nazionale, il ruolo di tutori del sereno e regolare svolgimento di ogni iniziativa pacifica,

per preservare l'ordine - per questione di ordine, per carità, perché nel 1936 c'era libertà di parola - uno striscione sul Duce sarebbe stato rimosso per motivi molto simili a quelli che lei ha illustrato adesso.

Visto che sono stati rimossi il questore e il Comandante dei carabinieri di Arezzo per non aver colpito con sufficiente durezza coloro che avevano il torto di contestare il ministro Boschi che era in visita in quella città (che peraltro è la sua), allora sarebbe forse stato il caso di assumere dei provvedimenti.

Alfano, alle organizzazioni internazionali che si occupano di diritti umani e di stabilire se l'attuale campagna referendaria è fatta come dovrebbe essere in un Paese democratico, oppure se ci troviamo già in un regime dittatoriale dove non si può dire: "Signor Presidente del Consiglio, lei ha fallito". Renzi, infatti, ha fallito

riferisco all'interrogazione con la quale la senatrice Taverna, unitamente ad altri colleghi senatori, chiede al ministro Franceschini notizie in merito all'inserimento del progetto relativo alla caserma Cerimant nell'elenco degli interventi per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, culturale, nell'ambito del piano «Turismo e cultura», da finanziarsi con l'assegnazione di un miliardo di euro a carico del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Al riguardo, la senatrice si richiama a un articolo comparso su «Il Fatto Quotidiano» del 6 maggio scorso, nel quale fra l'altro si faceva esplicito riferimento alla consorte del Ministro, aggiungendo che «non risulta agli interroganti che il Ministro o il consigliere, signora Di Biase, abbiano fatto smentita pubblica delle ricostruzioni giornalistiche». Si tratta di una asserzione non veritiera. Gli onorevoli interroganti hanno volutamente ignorato la puntale risposta del Ministro, pubblicata con adeguata evidenza dal medesimo quotidiano il giorno dopo e cioè il 7 maggio. Posso, quindi, limitarmi a richiamare quanto scritto dallo stesso Ministro e pubblicato dallo stesso quotidiano cui lei si riferisce e che leggo testualmente: «È vero. Tra i trentatré interventi finanziati con un miliardo di euro dal CIPE, uno dei più importanti, qualitativamente e quantitativamente, è il recupero della caserma Cerimant di Tor Sapienza. A fianco di progetti relativi a prestigiosi immobili dei centri storici, ve ne sono infatti alcuni che cercano di intervenire nella riqualificazione delle periferie urbane, vera sfida italiana dei prossimi anni e doveroso impegno per una cultura davvero progressista e di sinistra. In questo caso parliamo di un'area dismessa dell'esercito, collocata proprio in quella periferia romana che soltanto due anni fa fu teatro delle tensioni tra cittadini e immigrati e che diventerà un luogo per la cultura e la creatività, sul modello del famoso "104" realizzato nella periferia di Parigi. Vediamo secondo voi cosa avrebbe dovuto fare il CIPE: rinunciare a questa operazione, così concretamente e simbolicamente importante, perché fino a tre anni fa mia moglie, nata e cresciuta in un'altra periferia vicina a Tor Sapienza (l'Alessandrino), è stata, e da molto prima di conoscermi, consigliere municipale? dato che nel 2013 è stata eletta consigliere comunale, facendo diventare quindi il suo "feudo", secondo il vostro astuto modo di ragionare, l'intera Roma, avremmo dovuto rinunciare a finanziare anche la Galleria nazionale di arte moderna o Palazzo Barberini?! E per lo stesso motivo avremmo dovuto rinunciare a finanziare il completamento del Museo nazionale dell'ebraismo e della *Shoah* perché si trova nel mio "feudo" di Ferrara, o gli Uffizi perché nel "feudo" del Presidente del Consiglio o ancora i Musei Reali perché nel "feudo" di Fassino o Paestum perché in quello di De Luca e così via?».

di un sito che a nostro avviso poteva non avere la stessa importanza rispetto ad altre situazioni che erano state elencate, come ad esempio la pinacoteca di Brera, gli Uffizi di Firenze, Pompei (che cade a pezzi) o la Reggia di Caserta. Credo quindi che l'interrogante avesse tutto il diritto di sapere se rientrasse nel piano e se fosse così necessaria, vista anche la possibilità di essere indotti (in questo caso è capitato a a sospettare che il Ministro avesse destinato questi 40 milioni a una riqualificazione che a tutt'oggi non mi risulta essere cominciata e che sicuramente era di minore importanza rispetto ad altri progetti. Dico questo anche in relazione al fatto che ci fosse questa sospetta vicinanza con l'intenzione (potenzialmente meritoria) del Ministro di dedicarsi alle periferie, considerando anche che le periferie di Roma sono parecchie e non hanno avuto alcun tipo di attenzione quando

Signor Presidente, in riferimento all'interrogazione parlamentare in esame, si risponde sulla base degli elementi trasmessi dalla competente prefettura e da noi richiesti. In particolare, la stessa ha comunicato che il 4 gennaio 2016 la signora che indichiamo con le iniziali FL si presentava al pronto soccorso ostetrico dell'azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara e, dopo valutazioni, alle ore 00,43 del giorno 5 gennaio, veniva ammessa in reparto. Dalla relazione fatta pervenire dall'assessorato alle politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna per il tramite della suddetta prefettura, si evince che fu proposto alla signora di effettuare il travaglio in acqua: tale metodica viene proposta quale metodo naturale per contrastare il dolore, a detta dei sanitari coinvolti, e viene proposta anche in donne già instradate al percorso dell'analgesia epidurale. Dalla documentazione presente in cartella emerge che il travaglio è avvenuto in acqua. Per quanto concerne il presunto malposizionamento del feto al momento del parto, nonché la manovra di estrazione violenta che viene implicitamente ritenuta responsabile delle lesioni riscontrate sul bambino successivamente al parto, si precisa che dalla documentazione sanitaria - riferisce la Regione Emilia-Romagna - non risulta un malposizionamento del feto: in particolare, il bambino si è presentato al canale del parto in posizione cefalica che, a detta dei sanitari, non pare compatibile con il malposizionamento fetale. La documentazione (che (che la Regione ha visionato e ci ha trasmesso) rileva che il parto è stato spontaneo con presentazione di vertice OISA (che è la posizione corretta) con arto associato. La ricostruzione degli eventi, effettuata ancora una volta dal direttore sanitario in collaborazione con i sanitari della ostetricia, mette in luce che l'impegno della testa e del braccio sia stato risolto con una manovra di accompagnamento effettuata dal medico che assisteva il parto durante una contrazione. Risale, con elevata probabilità, a tale fase l'origine della frattura della clavicola, riscontrata successivamente attraverso controllo radiologico e non rilevata immediatamente, atteso che la stessa appariva in un primo momento composta. Non appaiono riferibili, invece, al periodo espulsivo le lesioni gastriche, spleniche e polmonari riscontrate dopo l'estubazione. La documentazione clinica dei primi minuti dopo il parto riporta un apgar al primo minuto di 8 e un apgar al quinto minuto di 10. Tale documentazione denota una transizione neonatale regolare. Il contenuto dell'interrogazione descrive le successive fasi dell'assistenza, evidenziando: la comparsa dei sintomi dell'emorragia digestiva (evento non fisiologico), l'aspirazione attraverso sondino nasogastrico e la somministrazione di antiemorragico, queste ultime sono procedure routinariamente eseguite nell'assistenza al al neonato fisiologico. Parimenti, il rigurgito di liquido amniotico, di colostro e di muco è da ritenersi tra gli eventi fisiologici. Si conferma, infine, che la somministrazione di antiemorragico è prassi nell'assistenza neonatale e, ad avviso dei medici, non va messa in relazione all'emorragia per ematemesi che fu riscontrata successivamente. La prima visita neonatologica, effettuata alle ore 16,15 del 05 gennaio 2016, evidenziava *facies* da stasi, che è un evento non eccezionale e transitorio nei parti vaginali (di cui, in genere, è prevista la regressione spontanea nelle successive 48 ore) e può verificarsi anche in assenza dell'impegno del braccio nel canale del parto. Dal diario infermieristico risultano, nella serata del 5 gennaio, "diversi rigurgiti di liquido amniotico, muco e colostro".

la stessa infermiera rilevava "vomito abbondante di sangue digerito e rosso vivo", per cui veniva allertato immediatamente il medico in servizio presso la terapia intensiva neonatale. Quest'ultimo, sopraggiunto quasi contestualmente alle ore 1,30 del 6 gennaio, effettuava gastrolusi e la valutazione clinica di ingresso in reparto per ematemesi. In questa occasione è stato fatto un prelievo per emocromo e coagulazione, i cui risultati, secondo questo diario, riportavano valori nella norma. Dopo alcune ore in cui il quadro clinico si manteneva stabile, al mattino il bambino riprendeva a sanguinare e, quindi, veniva chiesta la consulenza di chirurgia pediatrica e di endoscopia digestiva; venivano ripetuti gli esami ematologici che evidenziavano un'anemizzazione significativa ed esami radiologici che evidenziavano un pneumoperitoneo. Veniva praticata emotrasfusione di globuli rossi concentrati Dalla documentazione inviata dalla direzione sanitaria risulta essere stata effettuata l'esame specifico per indagare l'ematemesi. A seguito delle indagini clinico strumentali si poneva l'indicazione a un intervento chirurgico di laparotomia esplorativa che evidenziava una lesione

è stato in ventilazione assistita per 48 ore, con decorso del tutto regolare. Dopo l'estubazione, a distanza di circa 24 ore dalla documentazione clinica risultava un opacamento a carico del polmone di sinistra. Per questo motivo è stata chiesta l'esecuzione di un'endoscopia bronchiale che ha consentito la risoluzione del quadro atelettasico. In questa occasione, è stata anche rilevata la frattura composta della clavicola destra. Il piccolo MC, nato il 5 gennaio 2016, è stato dimesso a ventitré giorni di vita in buone condizioni generali. In data 22 gennaio 2016 la procura della Repubblica di Ferrara, presumibilmente su esposto-denuncia dei genitori FL e CV, ha chiesto l'acquisizione delle cartelle cliniche relative alla signora FL e al piccolo MC, che sono state consegnate. Successivamente, precisamente il 25 gennaio 2016, il pubblico ministero ha conferito incarico al medico legale, ai sensi dell'articolo 389 codice di procedura penale, di accertare eventuali responsabilità dei sanitari. L'indagine è ancora in corso.

il bambino ha superato la situazione, nonostante lesioni e cicatrici dovute anche agli interventi e a quanto

a mio avviso e ad avviso e delle persone che hanno vissuto questa esperienza, probabilmente si sono aggravati anche a causa della gestione dell'evento, per una somministrazione di farmaci e un succedersi di fatti che hanno probabilmente determinato una situazione di grave pericolo, anche di vita,

Anche la nascita in Italia è un problema sotto il profilo dei numeri e dal punto di vista sociale, dell'alloggio, delle tendenze demografiche; però, a volte, anche la gestione di questi reparti (quando non addirittura la loro soppressione in tante parti d'Italia, perché non c'è un numero di nascite che, secondo alcuni parametri, ne giustificherebbe la

sulla base degli elementi documentali che abbiamo chiesto e che ci ha fornito l'Agenzia italiana del farmaco. Prima di entrare nel merito delle altre questioni poste nelle interrogazioni, si forniscono alcune precisazioni con specifico riguardo all'allestimento, da parte dell'Aifa, di uno *stand* nell'ambito del «Meeting» di Rimini del movimento Comunione e Liberazione. A tale proposito, sembra opportuno precisare che questo tipo di allestimento dell'Aifa alla manifestazione fieristica «Meeting» di Rimini non è una novità, ma è risalente nel tempo. Infatti, vi ha già partecipato negli anni 2006, 2007 e 2008, al pari, peraltro, di altre amministrazioni pubbliche statali e locali che partecipano a quella iniziativa. Ed invero, l'Aifa riferisce che la scelta di allestire un proprio spazio espositivo nell'ambito della predetta manifestazione va inquadrata in una precisa politica investimento in attività di informazione e promozione, finalizzata a dare adeguatamente conto dell'impegno dell'Agenzia nel sistema sanitario del nostro Paese. Al fine di procedere a quell'allestimento, si è proceduto con regolare richiesta di acquisto all'ufficio affari amministrativi, contabilità e bilancio, motivata dalla circostanza

comunica che i vertici dell'Agenzia non sono iscritti, tantomeno militanti di Comunione e Liberazione. Passando poi alle specifiche domande degli onorevoli interroganti, si rappresenta che, quanto all'assunzione della dottoressa Caterina Latronico e del dottor Gianluca Polifrone, avvenute ad oltre un anno di distanza l'una dall'altra, con modalità e per profili professionali del tutto distinti, occorre rammentare che il consiglio di amministrazione dell'Aifa, con la delibera n. 36 del 14 ottobre 2014 (quindi due anni prima dell'assunzione del dottor Polifrone e ben distante anche dalla stipula della convenzione tra Aifa Consip, variamente commentata nelle due interrogazioni, avvenuta solo nel marzo 2015), aveva approvato un «progetto finalizzato allo sviluppo del Ruolo internazionale di Aifa ed allo svolgimento di nuove attività in ambito europeo ed internazionale», internazionale», prevedendo l'assunzione di tre unità da contrattualizzare a progetto per la durata di tre anni. Venivano quindi pubblicati, in data 15 gennaio 2015, l'avviso pubblico n. 15 e l'avviso pubblico n. 16, con cui, a seguito dell'esito negativo della ricognizione interna

a seguito della selezione condotta dalla commissione esaminatrice, presieduta dal responsabile delle relazioni internazionali (dottoressa Conti) e composta dal responsabile anticorruzione (dottor Di Giorgio) e dal responsabile dell'area legale (avvocato Mastroianni), venivano pubblicati gli esiti, individuandosi tre candidati, tra cui la dottoressa Caterina Latronico, come figure più qualificate a ricoprire tali posizioni. La dottoressa Latronico ha stipulato con l'Aifa un contratto a progetto della durata di tre anni, con un compenso lordo lordo annuo di 45.000 euro, quindi ben lontano dai 135.000 euro annui cui forse erroneamente si fa riferimento nell'interrogazione presentata dalla senatrice

possa rivestire, in forza del corrente rapporto di lavoro che la lega all'Aifa, alcun ruolo o funzione di tipo dirigenziale. Per quanto riguarda l'incarico conferito al dottor Polifrone di direttore della segreteria tecnica della direzione generale, è opportuno ricordare che l'attribuzione dello stesso è avvenuta sulla base di un avviso, pubblicato in data 19 aprile 2016, che non prevedeva come requisito di accesso il pregresso inquadramento in ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione. Il *curriculum vitae* del dottor Polifrone, allegato alla sua domanda di partecipazione alla procedura selettiva, delinea un profilo professionale qualificato per la posizione vacante e la scelta è avvenuta all'esito di una valutazione puntuale di tutte le candidature presentate e del conseguente giudizio tecnico, spettante all'amministrazione procedente, come comunica l'Aifa. L'incarico in questione, pertanto, è stato conferito sulla base di una valutazione tecnica discrezionale dell'Aifa, quale prerogativa tipica delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001

ai sensi del regolamento di organizzazione dell'Aifa, prevede competenze non scientifiche bensì amministrative, come dimostrano le precedenti assegnazioni dello stesso incarico. In merito In merito all'ipotizzata sussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 2013 «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico», a norma dell'articolo 1, 2012, n. 190, si precisa che l'Aifa, nel marzo del 2015, ha stipulato una convenzione per lo svolgimento di attività di supporto in tema di acquisizione di beni e servizi con la Consip SpA, ente di provenienza del dottor Polifrone. Il candidato, al quale è stato conferito l'incarico, non rivestiva all'interno della Consip SpA le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, né di amministratore delegato, né ricopriva le posizioni di dirigente, né svolgeva una stabile attività di consulenza a favore dell'Aifa, in quanto inquadrato nella Consip SpA come quadro/funzionario, con il ruolo di *account manager*. Un caso di inconferibilità dell'incarico al dottor Polifrone si sarebbe configurato solo se, nei due anni precedenti l'attribuzione dell'incarico di lavoro nell'Aifa, egli avesse ricoperto «le cariche di presidente con deleghe gestionali

attività di centrale di committenza per le pubbliche amministrazioni per cogliere l'obiettivo di razionalizzare la spesa. L'Agenzia sottolinea che aver espletato la gara con la Consip SpA ha prodotto, per in fase di stipula di contratto, un risparmio di oltre 1,2 milioni di euro (il vecchio contratto era superiore a 8 milioni di euro, il nuovo contratto è pari a 6.800.000 euro) senza considerare le diverse proroghe sul vecchio contratto, che hanno visto un impegno complessivo di spesa pari a 14 milioni di euro. il nuovo contratto stipulato tramite la Consip ha apportato all'Aifa significative migliorie in ambito informatico, in linea con l'Agenda digitale, quali: sistemi di pagamento;

infrastruttura per la dematerializzazione del processo gestione personale; utilizzo diffuso su tutto il personale della Carta nazionale dei servizi e firma digitale. È stato altresì avviato il sistema di monitoraggio dell'efficienza amministrativa dei centri per la sperimentazione clinica, all'interno dell'osservatorio, con geolocalizzazione e accesso all'intera documentazione degli stessi centri. In sintesi, la convenzione stipulata nella specie dall'Aifa con la Consip rappresenta un esempio positivo, in linea con la più recente legislazione in materia di accentramento degli acquisti finalizzata a realizzare politiche di *spending review* e nel contempo, di cogliere obiettivi di maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa. Quanto, poi, alla denuncia per danno erariale, cui viene fatto riferimento in una delle interrogazioni, l'Aifa riferisce che la stessa è scaturita da una missiva anonima

tra l'avviso per il conferimento dell'incarico contestato e la normativa sull'allargamento della pianta organica dell'Agenzia, che si pongono anzi in un rapporto di continuità logica e rispondono all'esigenza dell'Aifa di proseguire efficacemente nello svolgimento delle proprie attività, in attesa della finalizzazione delle procedure concorsuali previste dalla legge. Ciò risulta evidente dalla lettura dell'avviso per il conferimento di incarico pubblicato nel portale dell'Agenzia, che contiene esplicito riferimento alle disposizioni ora citate. La procedura per il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale dell'ufficio di segreteria tecnica della direzione generale si è svolta nella totale legittimità e nel pieno rispetto del principio di buon andamento dell'azione amministrativa. In particolare, sono state adottate modalità procedimentali idonee a garantire il trasparente e imparziale esercizio dell'attività amministrativa. Stante la necessità di coprire detto posto di funzione dirigenziale, caratterizzato da rilevanza strategica, anche in virtù della fase di riorganizzazione dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso. Poiché nessun dirigente dell'Agenzia ha presentato la propria disponibilità a ricoprire l'incarico, il direttore generale ha valutato le disponibilità presentate

in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi da conseguire e alla complessità della struttura interessata, degli elementi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in via prioritaria degli ulteriori requisiti, quali: «consolidata esperienza, almeno di 5 anni in uffici di diretta collaborazione»; «aver frequentato corso di formazione avente ad oggetto approfondimento del diritto costituzionale e del diritto comunitario»; «conoscenza dei sistemi informatici idonei all'espletamento delle funzioni»; «conoscenza della lingua inglese». Tali requisiti sono strettamente connessi alle funzioni dell'ufficio messo a interpello e sono rinvenibili nell'articolo 3, comma 1, lettera *a)* del previgente regolamento dell'Agenzia. In merito alla procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali, si evidenzia che la giurisprudenza ha affermato che la scelta di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, è orientata a ricercare non il migliore in assoluto, ma il soggetto in possesso delle attitudini necessarie per gestire, organizzare e dirigere il lavoro che afferisce all'incarico da ricoprire (si possono confrontare al riguardo la sentenza

al primo giudizio di inidoneità all'assunzione per un presunto *deficit* visivo, che pure viene citato nell'interrogazione, formulato dal medico competente in fase di visita preassuntiva nei confronti del dottor Polifrone,

dinanzi alla competente Azienda sanitaria che ha riconosciuto la piena idoneità del ricorrente, senza peraltro imporre alcuna prescrizione medica allo stesso. Per quanto attiene alla pubblicazione degli atti relativi al conferimento in oggetto, un altro punto sollecitato nell'interrogazione, l'Aifa riferisce di aver rispettato tutte le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, vigente all'atto del conferimento di quegli incarichi. In particolare, entro i tre mesi dal conferimento, l'Agenzia ha pubblicato nel proprio sito istituzionale: gli estremi dell'atto di conferimento, la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 39 del 2013, il *curriculum vitae* del dottor Polifrone e i relativi dati retributivi.

noi vogliamo Polifrone, ci inventiamo qualunque artifizio al fine di avere Polifrone, nonostante vi sia stata tutta una serie di violazioni (che comunque lei non mi ha chiarito). Le ribadisco infatti che sul sito dell'Aifa non sono state pubblicate né la determina del conferimento di incarico, ma solo i riferimenti, né il compenso stabilito a favore del Polifrone e che questa è una violazione dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2016. Così mi avete risposto. Quindi adesso dovrei prendere la risposta che lei mi ha dato,

scriverla. Signor Sottosegretario, non viene per niente evidenziato l'intreccio di relazioni e di favori intercorsi tra l'Aifa e la Consip, tra il dottor Pani e la famiglia Polifrone. Il Polifrone, assunto alla Consip dal 16 aprile 2013, diviene responsabile del procedimento relativo al bando di gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione, gestione, supporto specialistico, assistenza agli utenti e *hosting* del sistema informativo dell'Aifa, appalto dell'importo di oltre 11 milioni di euro, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 marzo 2015 (contratto stipulato il 20

Pochi mesi dopo, il 17 luglio 2015 veniva pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* il bando di gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di cassa dell'Aifa, che vedeva sempre il Polifrone quale responsabile del procedimento, con contratto stipulato il 1° aprile 2016. Il mese dopo, con determina del dottor Pani n. 664 del 6 maggio 2016, veniva assunto nell'Aifa anche il Polifrone, nonostante che fino

Sottosegretario, è avvenuto in palese violazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2013, che prevede l'inconferibilità dell'incarico a soggetti che «nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico». Il presidente dell'autorità nazionale anticorruzione Cantone ha recentemente denunciato, dietro al fenomeno della fuga di cervelli dall'Italia, una sorta di parentopoli nelle università. Chiedo con forza al Governo di agire contro la parentopoli nell'Aifa, che vede l'assunzione, oltre alla famiglia Polifrone, anche della compagna (madre di sua figlia) del dottor Pani, Valentina Mantua, denunciando questi episodi all'ANAC e alla procura della Repubblica. Signor Sottosegretario, la gestione di Aifa è positiva ed

perché hanno fatto un'altra delibera successiva rimpinguando ulteriormente il *budget* da dare a Comunione e Liberazione. Ma le sembra normale che il presidente dell'AIFA Melazzini, consigliere regionale lombardo, in sei mesi ottenga rimborsi per spese di quasi 100.000 euro? Le sembra normale che il dottor Pani, il direttore, abbia maggiori compensi per 700.000 euro e non li abbia ancora riversati? Ma le sembra normale tutto questo? Lei, signor Sottosegretario, deve dire

rese dall'amministratore delegato del gruppo ENEL, nell'ambito di un incontro svoltosi presso una struttura universitaria, non rientra nelle specifiche competenze del MISE, avendo tali dichiarazioni ad oggetto riflessioni personali sui criteri di organizzazione del lavoro aziendale e non coinvolgendo alcun aspetto di particolare competenza relativo al settore energetico.

che hanno ad oggetto un estratto delle dichiarazioni rilasciate dall'amministratore delegato del gruppo in data 14 aprile 2016, nel corso di un incontro con gli studenti dell'Università LUISS di Roma. È opportuno informare che, a seguito delle polemiche scaturite dalla pubblicazione delle dichiarazioni in parola, lo stesso amministratore delegato, rammaricandosi per le incomprensioni sorte, ha inteso chiarire il senso delle sue parole, presentando ufficialmente le proprie scuse ai dipendenti della sua azienda, evidenziando che le dichiarazioni, se estrapolate e non inquadrate nel contesto più circostanziato del suo intervento, anche se riferite in termini generali e non calate sul proprio ruolo nell'ENEL, si sono rivelate oggetto di uno spiacevole fraintendimento. L'amministratore delegato aveva invero già esposto, in occasione dello stesso incontro presso la LUISS, la propria visione del rapporto professionale e il proprio stile manageriale, improntato da sempre alla valorizzazione delle persone e alla promozione del benessere aziendale, definendo i collaboratori come fondamentali per il successo dell'azienda e sottolineando che è impossibile far carriera «tradendo, maltrattando, impaurendo e nascondendo i propri collaboratori; bisogna invece aiutarli, curarli e coltivarli tutti i giorni». A riprova di quanto sopra, la società ha comunicato i principali fattori rilevanti nella gestione delle risorse umane nel periodo coincidente con l'incarico dell'attuale amministratore delegato, evidenziando, in particolare, l'alto livello di partecipazione nelle relazioni collettive in un'azienda a partecipazione pubblica, la gestione del *turnover* senza ricorso ad ammortizzatori sociali e le modalità di inserimento in azienda attraverso un percorso di crescita e sviluppo nell'ambito dell'organizzazione aziendale, evitando il precariato, l'apertura e la trasparenza dei processi di valutazione dei comportamenti. Il gruppo ENEL ha infine reso noto di essere entrato nella Top 100 del nuovo indice di Thomson Reuters, che classifica oltre 5.000 aziende in termini di *performance* in materia di diversità e inclusione, mediante i dati ambientali, sociali e di *governance*, posizionandosi al venticinquesimo posto dell'indice, a testimonianza di come il gruppo abbia posto la non discriminazione, le pari opportunità e l'inclusione alla base della propria strategia industriale, elementi essenziali per il raggiungimento degli obiettivi più ambiziosi per una grande impresa.

il signor Starace ha risposto che per cambiare un'organizzazione aziendale è necessario che «un manipolo di cambiatori» che distrugga fisicamente i gangli che si oppongono al cambiamento; a tal fine bisogna «creare malessere» e poi colpire le persone che si oppongono al cambiamento. Non voglio continuare perché queste parole in italiano dicono una sola cosa. E vi dico di più: per quanto riguarda il sottoscritto, che il mondo del lavoro lo conosce, queste parole sono di una gravità inaudita. Se poi si

in un Paese democratico, ma se leggo che queste cose sono state fraintese o strumentalizzate, questi dubbi devono rimanere soprattutto al Governo perché ricordo che il lavoro è un diritto garantito dalla nostra Costituzione. Ripeto, se le scuse sono sincere, vanno accettate, ma non si permetta di dire che è stato frainteso o strumentalizzato perché l'intervento l'ho ascoltato per

alla mozione già approvata in Senato che chiede che per il settore risicolo sia garantita un'autonomia rispetto al meccanismo nazionale delle commissioni uniche nazionali (CUN), altrimenti il rischio reale sarebbe quello di mettere in difficoltà l'intera filiera risicola e le modalità di contrattazione che la caratterizzano.

maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare riguardano esclusivamente i soggetti interessati. Pertanto, in linea con gli impegni presi dal Governo, il settore risicolo può scegliere di avvalersi o no di tale strumento, cosa che ad oggi non è avvenuta. La costituzione di una CUN è subordinata alla richiesta della maggioranza delle associazioni di categoria del settore interessato che racchiude la volontà e l'accordo dei principali attori della filiera. L'eventuale successiva istituzione della CUN, tramite decreto ministeriale, si concretizza operativamente nella redazione di un regolamento di funzionamento che tiene conto delle peculiarità di ogni specifico settore.

ci soddisfa, ma staremo ovviamente attenti affinché venga rispettato il percorso definito, in quanto la concertazione, la definizione assieme alla filiera è fondamentale per la tutela e la garanzia che la nostra produzione nazionale di riso non abbia ulteriori danni rispetto alla concorrenza estera, che è molto aggressiva. Le CUN rischiano di essere altrimenti un vantaggio per la grande distribuzione, o meglio, i grandi produttori.

Come è noto certamente anche agli interroganti, l'attenzione del Governo sugli avvenimenti che hanno interessato e che interessano la ex Lucchini di Piombino è sempre stata e sarà massima. Il Governo, insieme alla Regione Toscana, ha messo infatti in atto un insieme di interventi per ridare a Piombino un ruolo importante nell'economia regionale e nazionale. La realizzazione del nuovo porto, insieme agli impegni per dare prospettiva all'attività siderurgica ed alle altre iniziative industriali quelle del gruppo Cevital con Aferpi) che si insedieranno nell'area liberata dall'altoforno, si ritiene ne siano la più chiara testimonianza. Nello specifico del piano industriale di Aferpi, non c'è dubbio che lo slittamento temporale rappresenti un problema da monitorare con la massima attenzione. Per questa ragione è stato chiesto all'azionista di Aferpi di accelerare la fase di progettazione e di costruzione dei nuovi impianti siderurgici, da realizzare con un piano finanziario che deve prevedere un impegno diretto importante dello stesso azionista. La risposta positiva di Cevital deve però completarsi con la disponibilità degli istituti di credito a supportare l'investimento che, si ricorda, supererà i 600 milioni di euro. La stessa attenzione è posta agli altri punti non meno importanti del piano industriale. Sia per le attività di logistica (in particolare nell'ambito delle disponibilità portuali createsi a Piombino con gli investimenti della Regione Toscana) sia per le cosiddette attività agroalimentari vi sono affidamenti e primi atti concreti: avvio delle fasi di progettazione ed acquisizione delle autorizzazioni propedeutiche all'esercizio di quelle attività. Per quanto riguarda le attività di bonifica, sono state completate tutte le fasi riguardanti l'approvazione dei piani presentati dall'azienda ed alle relative autorizzazioni sia nazionali (Ministero dell'ambiente e della tutela Risulta, inoltre, che sono stati emessi i primi bandi di gara per l'assegnazione dei lavori esecutivi. L'attenzione posta dalle autorità locali, oltre che dalle organizzazioni sindacali del territorio, è massima poiché l'avvio concreto dei lavori rappresenta un importante serbatoio che può ridurre l'impatto negativo determinato sulla occupazione dal ritardato avvio del programma di investimenti. Non vi è dubbio, infine, che la questione occupazionale rappresenti un fattore critico molto importante. Tuttavia si richiama il recente accordo firmato dalle organizzazioni sindacali territoriali e dalla direzione aziendale per l'inserimento con contratto di solidarietà, di tutti i lavoratori (oltre 800) che a novembre dovranno lasciare la Lucchini in amministrazione straordinaria. Per quanto riguarda la disponibilità di ammortizzatori sociali, si ricorda che la Aferpi rientra tra le aziende per le quali potrà essere utilizzata la cassa integrazione guadagni straordinaria fino al compimento del piano quadriennale e quindi fino a tutto l'anno 2018 in applicazione dell'articolo 42 del decreto legislativo del 2015, recanti disposizioni relative a trattamenti straordinari di integrazione salariale a seguito di accordi già stipulati (in vigore dall'8 ottobre 2016 quindi di recente). Su questa materia la sorveglianza del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sarà esercitata con il massimo rigore, anche oltre gli obblighi di legge che Aferpi deve rispettare. La migliore garanzia resta, in ogni caso, la quantità di investimenti che saranno effettuati entro i prossimi dodici-diciotto mesi e, in questo quadro, la quantità di risorse che Cevital dovrà mettere a disposizione per sostenere il piano nella sua interezza. Non c'è dubbio, infine, che gli impegni istituzionali per il miglioramento delle infrastrutture viarie (completamento della SS. 398 e del mancante raccordo ferroviario) rappresentano un aspetto decisivo per lo sviluppo dell'area piombinese, al di là della realizzazione dei nuovi impianti siderurgici. A tale proposito, sia il Ministero delle che i responsabili del gruppo Ferrovie dello Stato hanno dato garanzie che le due opere potranno essere completate nei tempi più rapidi, compatibilmente con l'effettiva disponibilità delle risorse già stanziate.

siamo in contatto con i lavoratori, quindi sappiamo quello che sta succedendo; farò quindi una sorta di resoconto di quanto è accaduto. A giugno 2015 c'era un accordo di programma presso il Ministero dello sviluppo economico con il gruppo algerino Aferpi che prevedeva la ristrutturazione dell'attività, con il passaggio dalla cokeria e altoforno alla fusione con forno elettrico; inoltre era prevista la bonifica ambientale dell'area industriale. Aferpi si era impegnata a investire 570 milioni di euro più altri 130 milioni (quindi 700 Poi, a giugno 2016, Aferpi ha presentato un altro progetto che, di fatto, stravolgeva quello precedente. L'accordo prevede un solo forno, anziché due, che invece di due tonnellate di acciaio ne produrrà solamente una.

Infine, ha proposto lo slittamento di due anni degli impegni assunti e questa è un'altra cosa molto preoccupante. È vero che i lavoratori sono stati chiamati dalla CIGS con i contratti di solidarietà,

quindi esserci la massima attenzione e, soprattutto, rispetto. Bisogna quindi verificare se questa ditta fornisce i requisiti giusti di affidabilità.